il Parlamento in seduta comune si riunirà nuovamente alle ore 18,30. La chiama avrà inizio dagli onorevoli senatori. In tal caso, la seduta della nostra Assemblea sarà organizzata per consentire ai colleghi di prendere parte alla votazione.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del Sud voterà a favore della proposta di risoluzione, anche perché non potrebbe essere diversamente, giacché le relazioni della Commissione antimafia vengono comunicate a entrambi i rami del Parlamento, ed entrambi i rami ne prendono atto e la fanno propria. «Zucchero non guasta bevanda», suol dirsi volgarmente: dunque può anche andare bene così. Mi fa particolare piacere la presenza e l'impegno del Governo per la soluzione delle problematiche poste poste in rilievo dalla Commissione antimafia, ma mi piacerebbe anche pensare che, così come avveniva nelle passate legislature, non vi sia la necessità di un dibattito in Parlamento e che dunque la forza politica della Commissione antimafia, che è stata sempre particolarmente forte e incisiva, possa far sì

Tuttavia ne abbiamo discusso, era utile discuterne e, probabilmente, se la discussione, piuttosto che sul documento, fosse stata sul fenomeno

Ho evidenziato anche talune lacune che sono certo i componenti della Commissione colmeranno in prosieguo di inchiesta; tuttavia, la possibilità di discutere su un fenomeno avrebbe potuto far sì che, invece di soffermarsi esclusivamente sul documento, di prenderne atto e di fare propri gli impegni del Governo, si cominciassero ad indagare le ragioni, la natura, le misure da adottare, pur in una situazione che vede la necessità per le casse dello Stato di fare ricorso alle lotterie e ai giochi e un'incapacità di controllo complessivo della vicenda. Se si Se si fosse arrivati a ciò, sicuramente il risultato sostanziale sarebbe stato di gran lunga superiore. Sono questi i dibattiti assolutamente auspicabili, che muovono certamente da una relazione, da dati che vengono acquisiti dai Ministeri, dalle amministrazioni autonome dello Stato e da tutte le fonti ufficiali, ma che devono spaziare in modo molto più ampio, al fine di costituire un momento di confronto su una visione sociale, politica ed economica di un fenomeno, di un problema e sulle possibili soluzioni per evitare quelle che sono certamente patologie

a qualcosa di più di una risoluzione che prende atto e impegna il Governo: addirittura ad una mozione condivisa, possibilmente all'unanimità, con un impegno politico e una forza incisiva di gran lunga superiore per il perseguimento di questi risultati. Tuttavia, è stato utile parlarne, ma il problema rimane: è un problema di particolare gravità, su cui comunque vanno accesi i riflettori e su cui l'attenzione delle stesse forze dell'ordine, della magistratura, ma anche, e soprattutto, in primo luogo, della politica deve essere ulteriormente incrementata. Quindi, plaudiamo all'operato della Commissione antimafia e ci auguriamo che, in prosieguo di stagione politica, si possa discutere nuovamente del fenomeno, su singole ipotesi relative a disegni di legge, ma che si possa al contempo ampliare il dibattito anche ad altra fenomenologia che comunque costituisce patologia della nostra società.

nel dire che dobbiamo riuscire a fare di più, nel senso che avendo ormai ben chiara la situazione (le relazioni della Commissione antimafia hanno messo insieme una serie di dati e di valutazioni che erano dispersi; il documento offerto è uno strumento di conoscenza dei diversi aspetti del problema, sicuramente non esaustivo, ma è uno strumento di conoscenza, di approfondimento e di intervento), è chiaro che dobbiamo agire. Non basta il voto che in questa sede ci accingiamo a dare, tutti d'accordo: proprio attraverso questa comune volontà politica noi dobbiamo fare altro. Vedete, quando abbiamo sentito al Comitato il rappresentante dell'Associazione concessionari apparecchi da intrattenimento, il dottor Giovanni Emilio Maggi, costui ha dichiarato «Abbiamo 350.000 apparecchi in rete e non c'è nulla di paragonabile al mondo. Le reti più grosse hanno 15.000-25.000 macchine e noi siamo a 15 volte tanto». il rappresentante dei concessionari sostiene che non è possibile che il nostro Paese si sia ridotto a tanto,

è stata che, essendoci i circuiti delle sale-tombola (e non si gioca con i fagioli, ma con i soldi), c'è spazio, perché vi è una rete fisica parallela che non è sotto controllo, e quindi bisogna contendere il terreno alla rete parallela.

quanto accaduto nell'ultimo anno, vale a dire il sequestro delle sale Bingo a Brescia, Cernusco sul Naviglio, Cologno Monzese, Cremona, Milano, Padova, Luca, Cassino, Ferentino, Sant'Arpino e Teverola, cioè proprio quei luoghi che dovrebbero essere tutelati e controllati. Insomma, l'organizzazione mafiosa pur non rinunziando alle tradizionali forme parassitarie di manifestazione, ossia l'imposizione del pizzo, nel settore del gioco e della raccolta delle scommesse su eventi sportivi sta cambiando volto nel senso che si sta strutturando sotto forma di imprese con connotati di normalità. La naturale conseguenza che ne deriva è che essendo notorio nel settore delle scommesse l'appartenenza di determinate imprese al circuito mafioso, rispetto al quale esse operano anche come lavanderia del denaro sporco, le altre imprese - quelle lecite e pulite - abbandonano quel tipo di mercato perché ritenuto non più conveniente e poco remunerativo.

Il Governo ha presente questa realtà, e l'impegno odierno è per noi importante.

un anno - dalla data di entrata in vigore di quella disposizione, linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia ludopatia conseguenti a gioco compulsivo. Ossia, è già malattia sociale riconosciuta, nel momento in cui in una legge si stabilisce che bisogna intervenire su questa malattia sociale che ha colpito oltre

La malattia è costo sociale ed economico: curare la malattia costa allo Stato e costerà molto di più di quanto lo Stato incassa attraverso la tassazione del gioco.

non debba portare a conseguenti determinazioni è una distrazione che non possiamo perdonarci. Noi abbiamo l'onere, il dovere di preoccuparci dei nostri concittadini; noi stiamo facendo il contrario, cioè stiamo assistendo alla crescita di un fenomeno che ha costi sociali con dazi criminali enormi. Dobbiamo fare il possibile per ridimensionare questo fenomeno distruttivo dell'economia della famiglia e così lucroso. La nuova frontiera d'interesse della criminalità organizzata ha preso il posto del traffico degli stupefacenti, essendo ormai a questi livelli. Questa è la realtà; quanto dobbiamo continuare ad urlare questa realtà se non si interviene? Per quante altre volte ancora

questa nostra disattenzione! Noi vi imploriamo: aiutiamo questo Paese disgraziato, il più appesantito da questo fenomeno al mondo!

credo che, anche ascoltando il fervore con cui i colleghi precedentemente si sono impegnati su questo argomento, si comprendano la gravità e la portata di questo triste fenomeno nel nostro Paese. Il Gruppo Lega Nord condivide appieno il sentimento di contrarietà per questa piaga della nostra società, che in maniera esponenziale si è amplificata proprio negli ultimi anni, arrivando a valori veramente notevoli: si parla di un volume d'affari

che lasciano il tempo che trovano, bisogna fare anche qualcosa di concreto: bisogna impegnarsi seriamente ed essere anche propositivi. Al riguardo, voglio sottolineare la recente proposta della Lega Nord di collegare la possibilità di accedere alle macchinette dei giochi *on line* con la tessera sanitaria. Questo ci permetterebbe anche di individuare, e possibilmente limitare, tutte quelle persone - purtroppo sono moltissime che si rovinano, giorno dopo giorno, su queste macchinette. Credo che bisogna essere costruttivi, al di là delle esternazioni demagogiche, pur sempre condivisibili perché sicuramente evidenziano la portata di questo problema; però, al di là delle proposte, tutti quanti

nell'obiettivo di ridurre questo triste fenomeno. Come sempre, quando vi è qualcosa di propositivo, la Lega Nord è a favore.

mi induce a svolgere una breve dichiarazione di voto sulla risoluzione promanante dai documenti dei senatori Li Gotti e Lauro, già approvati all'unanimità dalla Commissione parlamentare antimafia, che per il Partito Democratico è consapevolmente favorevole. Quelle relazioni - per la verità, molto puntuali ed allarmanti - necessitano non solo della condivisione di quest'Assemblea, ma anche di una sollecitazione ad ulteriori riflessioni sul piano della prevenzione generale, che devono necessariamente condurre ad un aggiornamento normativo coerente, non più eludibile. Invero già esistono al riguardo, proprio qui in Senato, disegni di legge che meritano un'accelerazione procedurale per meglio esaltare non solo i documenti esaminati, ma anche quella lungimirante legislazione antimafia a tutela delle fasce deboli di consumatori che, in un contesto socio-economico oltremodo fragile e compromesso, sono attratti da un miraggio propagandistico tra esasperante ed ipnotico. Mi riferisco, tra gli altri, ai disegni di legge nn. 2714, 2484 e 2909, rispettivamente a prima firma dei senatori Lauro, Li Gotti e - molto più modestamente - mia; essi spaziano dalla tutela dei minori alle misure antiriciclaggio, dalla trasparenza dei flussi finanziari alla modifica dell'articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, al divieto di pubblicità a tutela dei consumatori specialmente minori e fasce deboli. Tutto ciò premesso, nel confermare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico sulla proposta di risoluzione presentata, il mio intervento vuole essere anche un accorato appello, in sintonia con gli appassionati interventi dei senatori Li Gotti e Lauro, a declinare coerentemente questo dibattito calendarizzando rapidamente gli accennati disegni di legge.

e, dunque, dello sbarco del gioco d'azzardo legale nel tessuto socio-economico nazionale. Si è trattato di un evento inutilmente scongiurato da molti, giudicato inevitabile dai più; evento atteso, su fronti singolarmente opposti, assai fortemente dai soliti noti: da chi vi coniugava la prospettiva di enormi guadagni; da chi, forse un po' cinicamente, e soprattutto (così personalmente sostengo) in maniera assai miope, intravedeva qualche utilità per le casse dello Stato.

che dovrà condurci ad assistere al superamento del non virtuoso traguardo dei 70 miliardi di euro: un record europeo in termini assoluti; una delle prime posizioni, in termini proporzionali, a livello mondiale. Siamo tutti inevitabilmente orgogliosi dei primati del nostro Paese e ci piace che lo stesso primeggi in più campi. Il record dei 70 miliardi, per una popolazione adulta di una quarantina di milioni di persone, ce lo potevamo tuttavia francamente risparmiare.

nelle macchinette diffuse capillarmente negli esercizi pubblici di ogni città, di ogni paese: dal bar frequentato dal pensionato, al supermercato, punto di transito sostanzialmente obbligato per ogni famiglia italiana. miliardi di euro, in un anno, strumento di incomprensibile seduzione (per alcuni), di irresistibile seduzione per altri (sempre più per molti altri). miliardi di monetine da un euro - messe una accanto all'altra coprirebbero, se non sbaglio i conti, ben 7 milioni di chilometri, vale a dire quasi una ventina di volte la circonferenza del nostro pianeta destinati a traslocare dalle tasche di tantissimi nelle borse capienti ed ingorde di pochi biscazzieri, calati nel mondo della nostra impresa, all'apparenza giuridicamente legale - eticamente lascio a voi dire avendo a volte provenienze incerte e comunque normalmente e tendenzialmente da nessuno mai raccontate. Questi, dunque, i numeri principali della faccia legale di un fenomeno cui la Commissione bicamerale antimafia ha meritoriamente destinato plurime occasioni di indagine, in questa e in precedenti legislature, per determinare una sorta di campo base per l'esplorazione di quell'altra faccia che più pertinentemente le compete, che in verità non è solo quella del gioco illegale, ma è piuttosto quella della saldatura che il fenomeno del gioco - l'uno o l'altro gioco - determina con il mondo delle società criminali. Pensare che l'enorme quantità di danaro che transita nelle aree legali del gioco - per sapere a quanto ammonti il fatturato complessivo, comprendente anche le aree illegali, basta banalmente raddoppiare il dato, così come accertato dalle forze di polizia e dalla magistratura - lasciasse indifferenti le mafie sarebbe un'inescusabile ingenuità. Ed infatti non lo pensa nessuno, essendo anzi generalizzata convinzione dei più che tratti più o meno lunghi e più o meno decisivi (penso francamente, per quanto mi riguarda, che possano essere tranquillamente tolti i «meno» dalla i tratti più significativi delle filiere del gioco appartengano, in via diretta o indirettamente controllata, all'impresa mafiosa ovvero siano appannaggio - ma non cambia nulla - di imprese i cui capitali di avviamento altro non sono stati che l'espediente, per giunta assai proficuo, per la legalizzazione, la ripulitura dei proventi consueti dei traffici di mafia: gli stupefacenti, prima di tutto, ma non di meno la prostituzione, il saccheggio del territorio, i rifiuti e, da ultimo, il commercio dei migranti. Ma la commistione mafia e gioco - legale o illegale che sia - non si ferma purtroppo all'area intrinseca del gioco. Il guasto criminale - di quello sociale ed economico diversamente si dovrà dire si estende infatti a quei fenomeni di usura e di estorsione, per esempio, che costituiscono costanti accertate dalle forze di polizia nella massima parte dei luoghi dove il gioco è praticato. Anche qui, del resto, stupirebbe lo stupore di chi non vi ha pensato. Se infatti i casinò e le case da gioco da sempre vogliono dire, com'è a tutti noto, «cambia assegni» e «presta soldi», vale a dire qualcosa che praticamente nella quasi totalità dei casi potrebbe facilmente scambiarsi per usura, perché mai - più o meno in sedicesimo - ciò non dovrebbe essere in una sala Bingo o in un semplice bar, a monetine finite ? Tutto questo con il sovraccarico di sistematici fatti di estorsione e con la dovuta riflessione, che non è certo mancata alla Commissione antimafia, riguardo alle conseguenze che si determinano per via della frantumazione territoriale del fenomeno, alla luce di quella capillarietà di diffusione di cui prima dicevo, che è presupposto proprio per il controllo del territorio, cioè per la più antica e mai rinunciata ambizione mafiosa, presupposto di potere per la mafia e presupposto della maggiore e più cocente sconfitta per lo Stato legale, con quanto ancora ulteriormente ne segue e ne consegue, in termini di determinazione del mercato, per la collocazione degli ulteriori servizi criminali e di pervasività nella società. La Commissione antimafia e i deputati e i senatori che più si sono soffermati sulla questione - il senatore Raffaele Lauro, per tutti, nel Gruppo del Popolo della Libertà - non si sono tuttavia fermati all'esplorazione del solo relativo versante criminale. Sarebbe davvero pletorico, in questa sede, che si indugiasse nella parafrasi dell'efficace *report* che le relazioni di cui discutiamo rappresentano. Basta dire che il voto unanime dei componenti della Commissione la dice in sé lunga su quanto sia apparsa accurata, convincente e recante conclusioni non opinabili e non discutibili, l'analisi dei presupposti e delle conseguenze sociali che il fenomeno determina, gravando in maniera decisamente prevalente sulle fasce più povere della popolazione: un argomento che pure confina non trascurabilmente con l'*habitat* mafioso, che in tali contesti ha da sempre fabbricatola propria manovalanza. Cosa c'è di meglio di un drogato del gioco che, dopo aver perso tutto il frutto del proprio lavoro legale, altro non può fare che prestarsi allo straordinario illegale, per esempio ponendosi al servizio del mafioso di zona per rifornire i tossicodipendenti E' dunque un tratto, quello sociale, che deve far meditare tutti, addetti alla materia e non, per le molteplici implicazioni, dirette e proprie, e non, da cui è caratterizzato. Ed aggiungo infine l'ulteriore ed ultimo argomento su cui invito i colleghi e il rappresentante del Governo a qualche riflessione. Si dice, si è anche di recente affermato e stabilito in occasione delle ultime manovre finanziarie, che il fenomeno del gioco è utile alle casse dello Stato, perché determina ingressi erariali giudicati - sopratutto nell'emergenza - assolutamente essenziali. Si sono anche consumate polemiche in ordine alla correttezza o meno delle leve fiscali azionate e controllate (anzi in verità non molto controllate) nel settore. lo non voglio vestire panni che non mi sono propri, e - tra tutti - quelli dell'esperto di economia, ma non riesco francamente a fare a meno di pensare quale potrebbe essere la potenzialità di moltiplicatore industriale e commerciale dei 70 miliardi di euro, gettati nel gioco, gioco, ripartiti tra i vari attori del gioco, in minima parte riversati allo Stato, ove gli stessi fossero banalmente destinati al consumo, a qualsiasi consumo. È argomento posto, su cui non si riesce in verità ad avere risposta, quantomeno a puro livello argomentativo, e forse la ragione sta nei plurimi interessi che animano la questione: ho detto di quella dello Stato, del suo Ministero del tesoro; non si può certo tacere di quella della principale associazione di imprenditori, di quella Confindustria che non lesina quotidiane lezioncine di legalità e di antimafia e che pure contempla il gioco, quello legale, per carità, fra le proprie pieghe di associati. Ed allora occorre dire, non certo per consumare un esercizio di retorica che risulterebbe assai sciocco, che occorre davvero moltiplicare le riflessioni sull'argomento da parte della politica e di tutti quanti hanno responsabilità di governo e delle istituzioni, per virtuosamente orientare - ove possibile e ove lecito in una comunità che non può che continuare ad avere carattere liberale verso una cultura del positivo, che non è per nulla quella che appare dalle analisi svolte: meno ragionieri e più ragionamento, sia sul versante economico sia su quello sociale, e forse più risultati più positivi. Ho ascoltato le divergenti opinioni riguardanti la ritualità, o meno, della discussione che ha avuto oggi luogo, avente alla base documenti che già fanno parte del patrimonio di quest'Aula, alla luce dell'avvenuta loro approvazione da parte di un'articolazione parlamentare a conclusione di un processo costituzionalmente previsto tra le prerogative del Parlamento e stabilito con apposita legge. Altrettanto per quanto riguarda il voto della risoluzione che è stata presentata e che presto avrà luogo. Sono personalmente portato a credere che abbia ragione chi propende per l'irritualità dell'odierna iniziativa dell'Assemblea, e non già solo sotto il profilo formale, ma piuttosto per la non casualità che anche in questo caso contrassegna i contenuti delle nostre leggi e dei nostri Regolamenti. Si tratta tuttavia, per volerla mettere in termini positivi, di un'irritualità utile, probabilmente da non ripetere, ma senza dubbio oggi utile, perché ha condotto ad un pacato ma efficace *focus* su un tema che - senza dubbio di drammatizzazione - rappresenterà sempre più un problema, sotto i diversi profili che ho cercato di illuminare. I deputati e i senatori del Popolo della Libertà nella Commissione bicamerale antimafia hanno votato in maniera motivata e convinta le relazioni che sono oggi a presupposto della discussione. Altrettanto faranno, di qui a breve, per l'approvazione della proposta di risoluzione presentata, cosicché l'auspicabile sua unanime condivisione possa davvero rappresentare un'affermazione forte e conclusiva. *(Applausi dal

i rilievi svolti dal senatore Centaro, già presidente della Commissione antimafia nella XIV legislatura, e dal senatore Caruso, sono utili per precisare che l'odierno dibattito non può che svolgersi entro il perimetro normativo fissato dalla Costituzione, dal Regolamento e dalla legge istitutiva della stessa Commissione d'inchiesta, nel rispetto delle competenze e delle prerogative attribuite a ciascun organismo. L'Assemblea, in particolare, non si sostituisce all'attività d'inchiesta propria della Commissione antimafia ma, sulla base di quanto trasmesso al Senato dalla medesima Commissione e pubblicato in atti ufficiali, articola un dibattito secondo le modalità fissate dalla Conferenza dei Capigruppo, all'esito del quale non è preclusa la possibilità di esame e votazione di autonome risoluzioni, secondo la costante prassi regolamentare. A tale riguardo, ricordo che nel corso della XVI legislatura, Commissioni d'inchiesta monocamerali e bicamerali hanno presentato relazioni all'Assemblea sulla propria attività. In alcune occasioni si è dato corso anche a votazioni, uniformando così i lavori del Senato a quelli della Camera, dove già da tempo erano state ammesse votazioni su strumenti di indirizzo. Ricordo che la Camera dei deputati, nella seduta n. 419 del 18 gennaio 2011, ha votato risoluzioni connesse alla relazione territoriale della Commissione bicamerale d'inchiesta sui rifiuti; il Senato, nelle sedute n. 268 e n. 269

d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro; e infine, nella seduta n. 485 del 12 gennaio 2011, ha votato una risoluzione su un'ulteriore relazione intermedia

senatori. Dichiaro aperta la votazione. una nuova finestra"). Colleghi, vi informo che stanno assistendo ai nostri lavori gli studenti dell'Istituto aeronautico «Antonio Locatelli» di Bergamo, ai quali diamo il benvenuto.

Signora Presidente, signor Ministro, colleghi, questo è il momento (il primo, in cui il Senato della Repubblica è chiamato ad assumere responsabilità su un problema che oggi riguarda la condizione di vita di almeno un milione di italiani: la malattia di Alzheimer, la demenza, il deterioramento cognitivo.

Abbiamo presentato la mozione n. 320 un anno fa, nei giorni in cui si celebrava la XVII Giornata mondiale dell'Alzheimer, istituita dall'Organizzazione mondiale della sanità e dall'*Alzheimer's Desease International* la esaminiamo oggi alcuni giorni dopo la celebrazione della XVIII Giornata, il 21 settembre scorso. Noi siamo qui in rappresentanza del popolo per affrontare i problemi del nostro Paese, per conoscerli, per approfondirli, per decidere, in questo caso per indirizzare le politiche del Governo e delle Regioni e i servizi degli enti locali e del Servizio sanitario nazionale, per sostenere le famiglie, le associazioni e il volontariato che sono sulla frontiera, cito per tutte per investire fortemente nella ricerca, per sensibilizzare adulti, giovani e anziani su un problema che incide sulla vita di molte persone e di molte famiglie, che preoccupa l'opinione pubblica e che ancora non è adeguatamente esplorato, un problema sicuro nel futuro, l'epidemia silente del terzo millennio, una grande patologia sociale. Colleghi, a che punto siamo? L'ampiezza del fenomeno è descritta dai dati. International* (ADI) si parla di 36 milioni di malati nel mondo, di cui 6 milioni in Europa e un milione in Italia. Le demenze sono destinate ad aumentare fino a raddoppiare nei prossimi vent'anni, con un incremento di 150.000 nuovi casi all'anno in Italia; 27 milioni di malati nel mondo non ricevono, né diagnosi, né cure, né informazioni, né trattamento. Una malattia che non di rado è vissuta nella solitudine e nell'abbandono

È una patologia che costa, non solo sul piano sanitario ma economico e sociale. È stata elaborata la Carta dei diritti dei malati di Alzheimer, che ha posto correttamente il problema nel quadro dei diritti costituzionali. Sono cittadini cui è dovuta la cura. Vi sono in Italia molteplici esperienze sul piano sanitario e sociale, pur in un quadro di disomogeneità sul territorio nazionale, che ci consegnano ormai livelli maturi e consolidati. Non siamo cioè agli inizi della conoscenza del fenomeno; sappiamo ormai che è importantissima la diagnosi precoce: questa è la nuova sfida e deve essere affrontata in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Sappiamo che la prevenzione è fondamentale, che si possono individuare i soggetti a rischio, che solo attraverso l'osservazione ma anche attraverso test e *marker* biotecnologici, quindi osservazione più esami, come avviene in Francia dove sono stati scoperti test specifici non costosi determinando uno *screening* assai utile, così come assai utile è l'attività fisica e mentale. Sappiamo che si devono preparare sia medici di base che personale qualificato, che la prevenzione consente di evitare terapie errate, con conseguente risparmio di energie e costi. Sappiamo che l'incidenza sociale della malattia impone la ricostituzione del fondo per la non autosufficienza, ora azzerato. Negli anni precedenti il fondo ha consentito, con una quota mirata, interventi di sostegno alle famiglie, gruppi di mutuo aiuto, centri diurni specializzati, ricoveri di sostegno e sollievo. All'INPS ora raccomandiamo grande attenzione nella verifica delle condizioni per il riconoscimento dell'invalidità e per l'assegno di accompagnamento, perché in questi casi davvero l'apparenza può ingannare. Sul piano sanitario si deve considerare la necessità che siano autorizzati farmaci specifici, non con tabelle impositive ma secondo i soggetti, la loro concreta condizione e la relazione terapeutica con i medici. Grande attenzione e investimenti devono essere dedicati alla ricerca, il motore di ogni avanzamento terapeutico, ma è la solidarietà dell'intera società, della città, della comunità che deve essere evocata. Vi sono esperienze consolidate e innovative che devono essere riconosciute come buone pratiche perché hanno conseguito buoni risultati, perché il buon accompagnamento della malattia è parte della cura. Io conosco le esperienze della mia terra, di Parma e Reggio Emilia, del "Caffè Alzheimer" di Pavullo nel modenese, aperto agli anziani affetti da demenza, ai loro familiari e ai cittadini. Conosco l'esperienza dell'Emilia-Romagna che da 11 anni ha attivato ambulatori sul territorio mettendo in rete gli interventi e i soggetti competenti sul piano della diagnosi, della presa in carico del sostegno alle famiglie, dei servizi territoriali, sanitari e sociali, delle aziende sanitarie, dei medici di medicina generale e degli specialisti. Poiché oltre la metà dei problemi di demenza sono presenti nelle case protette, si è avviata la formazione degli operatori, mentre è assai attiva la collaborazione con le diverse espressioni associative del volontariato. Presidente, la mozione impegna il Governo a conseguire alcuni essenziali obiettivi: ad operare una sorta di censimento su tutto il territorio nazionale; a dare vita a un osservatorio nazionale con un tavolo di lavoro che metta in luce problemi e soluzioni costituendo un forte punto di riferimento nazionale per la rete; ad emanare linee guida per tutto il territorio nazionale; a promuovere la ricerca in collaborazione con istituti, centri di ricerca, università; a impegnare le Regioni in politiche sanitarie che sostengono le famiglie attraverso i servizi sanitari e sociali; a promuovere la formazione dei medici di base, di tutti gli operatori, comprese le cosiddette badanti; a ripristinare il fondo per la non autosufficienza con risorse mirate agli interventi in materia - i fondi per le persone più deboli sono davvero prioritari - e a sostenere le famiglie e le associazioni di volontariato così attive sul territorio. Signora Presidente, la crisi economica e la scarsità di risorse aumentano la paura che le persone più deboli siano abbandonate al loro destino. Non può essere così: l'Italia può essere ancora, come è stata, all'avanguardia in Europa nell'esperienza del sociale, del *welfare* e dell'educazione. Sono certa che il dibattito in Aula arricchirà le nostre riflessioni, ma soprattutto stimolerà tutti (Parlamento, Governo, istituzioni, servizi, volontariato sociale e ricerca) a interventi concreti per migliorare lo stato delle cose dando speranza a chi oggi combatte la sua più grande personale battaglia e fiducia nel futuro all'intera società. Penso che vinceremo questa sfida se potremo contare sull'impegno delle pubbliche istituzioni e, insieme, sulla coscienza solidale dell'intera società italiana.

*(IdV)*. Signora Presidente, la malattia dell'Alzheimer è diventata il terzo problema sanitario dopo le malattie cardiache, polmonari e tumorali. Solo in Italia ogni anno si registrano 150.000 nuovi casi di persone ammalatesi di Alzheimer. In occasione della giornata nazionale, come ha ricordato la collega, celebrata il 21 settembre, International* (ADI), l'organizzazione che lavora in tutto il mondo per migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da questa malattia e delle persone che li assistono, comunica i dati del proprio rapporto mondiale sulla malattia. Nel 2009 l'ADI stimava in 36 milioni la popolazione mondiale affetta da questa malattia e prevedeva il raddoppio di questa cifra Nel 2010 veniva evidenziato come la spesa mondiale per la cura ammontasse a più dell'1 per cento del PIL globale e che, se la spesa fosse un bilancio nazionale, sarebbe stata pari a quella del diciottesimo Paese più ricco del mondo. Immaginate, colleghi, quanto costa questa malattia. La diagnosi tempestiva

Sfortunatamente, ancora grandi ostacoli si frappongono all'accesso alle cure: ci sono veri e propri pregiudizi ancora troppo diffusi e purtroppo anche nei Paesi con buone risorse, con un buon livello di informazione ed alto reddito. Tuttavia, i fatti e le raccomandazioni esposti nel rapporto ADI e in numerose altre pubblicazioni, se presi in considerazione, sono in grado di sollevare i veli dalla malattia e preparare la strada ad un trattamento e ad una cura grandemente intensificati. Ogni persona affetta da tale malattia ha diritto ad una diagnosi tempestiva. L'intervento deve essere assicurato fin dal primo momento, quello in cui il malato e i suoi familiari per la prima volta prendono coscienza della malattia e sono costretti a confrontarsi con essa.

di prendere parte quanto più possibile alla pianificazione della loro vita dopo la diagnosi, e di assumere importanti decisioni circa i futuri trattamenti e cure. Essa permette l'accesso al percorso di trattamento, cura e supporto basati sull'evidenza, durante il decorso della malattia. L'impatto di una diagnosi di Alzheimer dipende in massimo grado da come è fatta e comunicata. Quando i soggetti affetti e i loro familiari vengono ben preparati e supportati, i sentimenti iniziali di *shock*, rabbia e dolore vengono controbilanciati da un senso di rassicurazione e di possibilità di controllo. La diagnosi tempestiva - lo dico a quei colleghi

Soltanto attraverso l'acquisizione di una diagnosi essi possono avere accesso ai farmaci disponibili e alle terapie non farmacologiche che potrebbero migliorare il loro stato cognitivo ed elevare la loro qualità di vita. Come abbiamo scritto tra gli impegni di questa nostra mozione, l'aumento della possibilità di diagnosi precoce può essere ottenuto mediante programmi di educazione ad indirizzo pratico rivolti ai medici di base, l'introduzione di servizi accessibili di diagnosi e cura degli stadi iniziali della malattia, la promozione di un'efficace interazione tra le diverse componenti del sistema sanitario. sanitario. In Italia le risposte ai bisogni dei malati e di chi li assiste risultano essere ad oggi scarse e disomogenee. L'80 per cento dei malati è assistito unicamente dalla famiglia e la durata della malattia è compresa tra i sette e i dieci anni dal momento della diagnosi. è un ostacolo che si oppone significativamente al miglioramento della qualità di vita dei soggetti affetti da Alzheimer o da altre tipi di malattie analoghe, dei loro familiari e di chi li assiste. Cure mediche e altri interventi di supporto sono disponibili solo per i soggetti che hanno cercato e ricevuto una diagnosi. Ad esempio, i trattamenti farmacologici e gli interventi psicologici e psicosociali attualmente disponibili possono essere efficaci, negli stadi negli stadi iniziali della malattia, nel migliorare i sintomi dei pazienti affetti da demenza e nel ridurre lo stress di chi li assiste. È a tal fine che si chiede un maggior impegno sul fronte della ricerca. Non dimentichiamo

e che, se applicati precocemente nel corso della malattia possono risultare più efficaci nel permettergli di continuare l'opera di assistenza a casa, evitando o ritardando in tal modo l'istituzionalizzazione Intensificare l'uso degli attuali trattamenti basati sull'evidenza, in particolare di quelli applicati negli stadi iniziali della malattia, permetterebbe ai sistemi sanitari di prepararsi meglio ad adottare nuove tecnologie Infine, nell'insieme, i rapporti dell'ADI hanno dimostrato chiaramente come l'Alzheimer costituisca anche uno dei più significativi problemi economici, oltre che socio-sanitari. il costo sociale annuo per ogni paziente affetto da demenza ammonta mediamente a circa 24.000 euro. In Italia il costo sanitario annuo varia,

Se anche a questa cifra si sommassero i costi per gli interventi precoci, il risparmio netto che si otterrebbe ritardando l'istituzionalizzazione del paziente sarebbe di più di 7.000 euro per soggetto durante il decorso della malattia. Il miglioramento della salute e della qualità di vita di chi assiste, oltre che del malato, rende questo investimento ancor più conveniente: si potrebbero realizzare importanti risparmi in un momento in cui i Governi sono molto preoccupati per l'aumento dei costi sociosanitari; secondo

si perde la memoria: non solo la memoria dei ricordi, ma anche quella dell'identità. Chi ne è affetto muore ancor prima di morire. Questa è una malattia che per l'uomo è un po' come il virus per un computer: entra e non cancella solo i *record,* ne distrugge anche l'identità e blocca il sistema. Il sistema "uomo malato di Alzheimer" (questo è il nome della malattia) smette di compiere le operazioni che prima venivano venivano svolte automaticamente. Fu chiamata Alzheimer dal nome dello scienziato che tra i primi si dedicò allo studio della proteina, che si chiama beta-amiloide, che è al centro delle discrasie, delle disfunzioni dei meccanismi che rendono impossibile la comunicazione fra le varie cellule nervose. Ma vi è anche un altro nome per identificare questa che è tra le patologie della demenza la più devastante, la più rilevante. Il nome è «malattia delle

il quadro patologico che accompagna la vita di queste persone sventurate: amnesia, che è la perdita della memoria di sé; afasia, che è l'impossibilità di comunicare tramite il linguaggio verbale con altre persone; agnosia, che non permette di riconoscere luoghi, persone, cose, anche se si tratta di luoghi, persone e cose entrati da sempre da sempre e per sempre nella quotidianità della vita; infine, aprassia, che è l'incapacità, prima parziale e poi progressivamente totale, di compiere anche le più elementari operazioni, determinando un blocco del sistema che regola i movimenti volontari, come quello più banale di vestirsi al mattino. Di questo ci stiamo occupando: si tratta di una malattia che affligge 35 milioni di persone nel mondo, che interessa oltre 600.000 persone nel nostro Paese e che vede, per i dati modesti di cui disponiamo, un'incidenza nella popolazione variabile

la terza età, ma che non esclude e non risparmia le persone che sono addirittura in età produttiva, ovvero quelle con meno di 65 anni, che vengono improvvisamente strappate alla loro vita di relazione e alla loro attività produttiva, determinando conseguentemente l'inesorabile tragedia legata al reddito e al sostentamento del nucleo familiare.

una progressiva attenzione, che ha portato l'Organizzazione mondiale della sanità a stabilire che la patologia dell'Alzheimer è una priorità nell'agenda internazionale, Non c'è patologia, non c'è malattia che non determini una sofferenza psichica, oltre che fisica. Ciò accade per le patologie neoplastiche, che determinano

esame ha però una ricaduta e un impatto sociale assolutamente enorme e inquietante, perché investe senz'altro il paziente che ne è affetto, ma investe in pieno e coinvolge anche il nucleo familiare, che rappresenta il primo riferimento, la prima rete di protezione sociale che si offre come risposta immediata alla solitudine e all'inquietudine di chi è improvvisamente morto alla vita, ancor prima che lo stabilisca il medico con l'apposito certificato.

dei bilanci pubblici - che hanno consentito di dare una risposta, che non riguarda soltanto l'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza sul versante dei servizi socio-sanitari e assistenziali, ma è anche una risposta che declina in modo profondo e pieno quei principi di universalità, di solidarietà, che ispirano la politica sanitaria del nostro Paese e che dobbiamo tutelare, probabilmente riproponendo al dibattito dell'Assemblea il tema del cosiddetto *welfare* selettivo, prima che il sistema imploda, all'interno di un patto intergenerazionale che, anche per le dinamiche anagrafiche, rischia di far saltare il banco. Signor Ministro, noi abbiamo seguito, e anche con attenzione, quanto sino ad oggi è stato fatto. Il Piano nazionale della prevenzione 2010-2012, che mi pare sia oggi all'attenzione della Conferenza permanente Stato-Regioni, prevede espressamente la necessità di dare una risposta alla prima esigenza, che è quella del governo clinico complessivo delle demenze, che sia in grado di utilizzare nella pratica clinica le evidenze scientifiche,

coordinamento delle attività dei diversi servizi dedicati e il fronte dei diversi operatori socio-sanitari, dai medici di medicina generale ai familiari a tutti i decisori, ivi comprese le associazioni di volontariato, che - lo dico con una nota di plauso particolare - svolgono un'attività che non di rado vicaria anche la carenza dell'offerta del Servizio Abbiamo visto lo schema di decreto con il quale vengono revisionati i LEA e abbiamo letto con apprezzamento, signor Ministro, che lì c'è scritto qualcosa sulla necessità e sulla previsione concreta di attivare servizi, nuclei, realtà residenziali e semiresidenziali dedicati alle persone con demenza, con specifiche garanzie per il sostegno e il potenziamento dei servizi erogati, ivi compresi gli interventi di sollievo.

all'attenzione del presidente Tomassini e dell'intera Commissione, per il previsto parere. Lì c'è un riferimento alle strutture extraospedaliere chiamate a rispondere ai bisogni socio-sanitari dei pazienti con appositi nuclei specializzati, i cosiddetti nuclei Alzheimer per la diagnosi precoce; vi sia anche, con le misure già previste dal decreto del 29 novembre 2001, l'erogazione a carico del Servizio sanitario delle prestazioni di assistenza domiciliare integrata, attraverso provvedimenti di esenzione dal pagamento dei *ticket* per l'assistenza farmaceutica. Tuttavia, riteniamo che ancora qualcosa debba essere fatto.

indicato delle cifre: quanto può costare l'Alzheimer; quanto costano le malattie della demenza; quanti sono i pazienti; come sono distribuiti sul territorio; come i territori, nell'ambito del nostro Paese, da Regione a Regione, rispondono rispetto all'esigenza dei pazienti. Questo lo sappiamo: c'è una differenza talvolta talvolta molto ampia fra Regione e Regione e c'è la necessità di creare un livello di maggiore omogeneità

esigenza, che interpella non soltanto la scienza e gli operatori sanitari, ma anche le coscienze di ciascuno per le implicazioni cui ho fatto poc'anzi riferimento. quanto sia necessaria la formazione per il personale, perché nella sanità il patrimonio dei saperi scade del 50 per cento ogni otto anni. I percorsi di formazione continua per i medici e per tutti gli operatori della sanità rappresentano un obbligo già previsto dalla legge, che ci suggerisce evidentemente di individuare, all'interno dei programmi dell'educazione continua in medicina, specifiche sessioni destinate all'approfondimento e all'aggiornamento su questa materia. Quanto alla ricerca, indubbiamente oggi la risposta è ancora molto parziale. La terapia farmacologica può intervenire sui sintomi, ma non sulle cause. Quindi oggi non si può che intervenire mitigando gli effetti devastanti di questa patologia. La ricerca rappresenta quella fiammella accesa che resta il punto di riferimento per una comunità che con il fiato sospeso segue i destini di un paziente destinato all'oblio e molto indifferenza da parte della realtà dove egli vive. È necessario, signor Ministro, che le cose buone che sono state scritte e l'attenzione che il Governo ha dedicato a questi capitoli capitoli trovino il più immediato riscontro. Per questo ritengo necessarie che venga, nei tempi più brevi, definita non soltanto la procedura per l'approvazione del Piano sanitario, ma anche la promozione delle linee guida per la prevenzione, per la prevenzione, la diagnosi precoce ed il trattamento dei pazienti affetti dal morbo di Alzheimer al fine di ottenere una condizione adeguata per una programmazione, una pianificazione e per l'allocazione delle risorse economiche là dove servono e per le finalità per le quali servono, all'interno di una regia complessiva che non può che essere nazionale, coordinata, naturalmente, a livello territoriale, nel rispetto delle competenze delle Regioni. di individuare ogni iniziativa utile a far lievitare il senso di partecipazione, di consapevolezza, di educazione sanitaria dell'intera comunità, affinché questa possa affrontare con maggiore certezza

una prerogativa dell'uomo fino a quando non esala l'ultimo respiro. Io credo che anche la sollecitazione derivante da queste mozioni, dal dibattito sviluppatosi, il profondo

unitamente al Governo, una risposta più adeguata ad una domanda che merita di essere completa rispetto all'esigenza crescente e alle prospettive di una patologia la cui incidenza, è destinata ad aumentare in modo esponenziale, con costi enormi. Tali costi possono essere governati e contenuti anche favorendo la diagnosi precoce e con la pronta risposta a tutte quelle richieste che il mondo della sanità elabora e che lo stesso mondo dei pazienti, tramite le rispettive associazioni, da tempo ha presentato in tutti convegni e nelle giornate dedicate all'approfondimento del tema. *(Applausi dal Gruppo*

che praticamente, a causa anche dell'esperienza che ormai si ha nel mondo e in Italia, vengono riferiti dati e vengono fatte proposte che sono del tutto condivisibili (e sono sicura che non sarà lei

per chi ha un malato di Alzheimer in casa il tempo non si definisce, perché a causa della notte che cade sul cervello del malato-parente il buio arriva per tutta la famiglia. All'inizio non ci si rassegna nemmeno quando si vedono i primi sintomi di chi non ti riconosce più, di chi non riconosce il luogo in cui si trova, di chi non sa vestirsi o mette dei vestiti sbagliati. Anche la persona interessata, più è colta e più ha avuto un cervello attivo, meno si adatta a capire che cosa le sta accadendo.

medici (sa che io ho una solidarietà speciale per i nostri medici di medicina generale) siano esperti: non tutti sono neurologi, non sono tutti psichiatri, non sono tutti psicogeriatri. Quindi, si fa fatica ad avere una diagnosi precoce dell'Alzheimer o di una demenza senile. Pertanto credo di poterle chiedere, ad integrazione di tutti i suggerimenti delle nostre mozioni, di ricordarsi che strumento essenziale è l'UVA, l'unità di valutazione Alzheimer. Lei sa che sono solo 500 in Italia, a fronte di un milione di malati acclarati, e l'UVA è un sistema nel quale gli operatori più avvertiti - perché quello studiano: parlo di neurologi, psichiatri, geriatri, con anche altre figure come gli infermieri - riescono a dire e a dare anche al medico della famiglia e ai familiari suggerimenti opportuni. Abbiamo sentito evocare il fatto che non sempre sono a disposizione i farmaci. I farmaci forse sono a disposizione; il problema è la corretta somministrazione, come dosaggio, oltre che come qualità. Quindi, occorre che ci sia alla base il suggerimento di chi

non di una patologia, ma di quelle relazioni umane, affettive, che si interrompono o diventano alterate. Quindi, il malato deve essere inserito in una rete protettiva sia sanitaria, per i suoi bisogni di di malato, sia sociale, perché rimane un cittadino. Signor Ministro, credo che in quest'Aula, anche con un po' di commozione, possiamo ricordarci che questi malati rimangono cittadini.

Abbiamo bisogno di far sapere che, quando si è deboli, lo Stato c'è, anche a fronte del regionalismo che non solo non denunciamo, ma apprezziamo; alcune malattie, però, devono essere messe in carico all'intera Nazione.

Ministro, onorevoli colleghi, non ho bisogno di dilungarmi perché c'è più partecipazione di quanto crediamo su tale argomento.

vi è ancora spazio per fare selezione per ciò che serve davvero, per ciò che serve di meno e per ciò che non serve affatto, e nel campo diagnostico e terapeutico, soprattutto attraverso i farmaci, di spazio ce n'è tanto. *(Applausi

oltre che nell'età anziana, anche abbastanza precocemente: capiamo bene che è tanto più devastante quanto più giovane è l'età di insorgenza della patologia.

laddove si riescano ad individuare precocemente i sintomi del cosiddetto deterioramento, purtroppo non si possono applicare protocolli di terapia specifici, come sanno benissimo

individuate ad oggi le caratteristiche eziopatogenetiche, non esiste una terapia specifica, per cui la precocità della diagnosi non serve ad aiutare di più l'ammalato. Quello che può essere più utile in questo momento è non distrarre l'attenzione

i soggetti affetti da malattia di Alzheimer hanno la possibilità di accedere all'invalidità civile, quindi all'indennità di accompagnamento, anche se sappiamo tutti benissimo a quanto ammonta il beneficio economico:

infatti la conoscenza della vera incidenza della patologia, ma considerato comunque che statisticamente, anno per anno, la percentuale di questi malati tende ad aumentare, è chiaro che è una esigenza

importantissimo quello che ha detto la senatrice Garavaglia sull'unità di valutazione Alzheimer: la diagnosi precoce e appropriata è fondamentale e deve essere fatta da ambienti specialistici, che si stanno purtroppo riducendo dopo la fine della sperimentazione. incentivare la terapia e la ricerca, perché purtroppo la malattia di Alzheimer sappiamo essere poco redditizia per le strutture che erogano sanità e molto costosa per i farmaci. La

perché il malato di Alzheimer finisce di essere un problema sanitario e diventa un problema assistenziale: questo non è assolutamente accettabile. Non tutte le situazioni sono rosee come quella dipinta dal film di Pupi Avati «Una sconfinata giovinezza», dove il tema è trattato in modo molto delicato ma anche molto edulcorato. Purtroppo il problema è sulle spalle di molte famiglie. Quindi il tema della rete dell'assistenza e di spostare soldi dall'acuzie alla cronicità è fondamentale per il sistema sanitario nazionale e per i sistemi sanitari regionali. Questo è il terzo punto che volevo sottolineare.

tutte le richieste presenti nelle mozioni: interventi e misure di politica sanitaria, mappe aggiornate; ottimizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici con la riorganizzazione e il potenziamento delle UVA;

verifica dell'attività; istituzione di una funzione di coordinamento permanente per le demenze. Il Governo è dunque impegnato in questo senso, e vorrei garantire alla senatrice Mariapia Garavaglia che effettivamente questo documento sarà oggetto di un accordo Stato-Regioni in cui si impegneranno le Regioni a trovare, nell'ambito del Fondo sanitario nazionale, le risorse necessarie per questo tipo di attività.

non mi posso impegnare in questa sede a trovare nuovi stanziamenti, ma sicuramente a trovare risorse per le demenze in quelle attualmente disponibili. Questo è l'impegno che posso prendere. Procedo quindi a leggere le riformulazioni